Onorevoli colleghi, come è ormai tristemente noto a tutti voi, nella mattinata di ieri un ordigno fatto esplodere al passaggio di un convoglio militare nella provincia di Herat, in Afghanistan, ha provocato la morte di due soldati italiani, due alpini della Brigata Taurinense: il sergente Massimiliano Ramadù e il caporalmaggiore Luigi Pascazio. Ancora una volta l'Italia piange due suoi giovani figli caduti per la pace, due soldati impegnati a consolidare la democrazia e la stabilità dell'Afghanistan e, con esse, la sicurezza e la libertà di tutto il mondo dalla piaga oscura del terrorismo. Non dobbiamo dimenticare mai che è la difesa di questi irrinunciabili valori a motivare ogni giorno la permanenza in quella terra difficile, martoriata da anni di guerre e di violenze, di una Forza di pace internazionale in grado di accompagnare il popolo afgano nel difficile cammino verso il rafforzamento della democrazia, dell'indipendenza e della sicurezza all'interno dei propri confini. Sono certo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea nel rivolgere un pensiero di profondo cordoglio e di commossa partecipazione al dolore delle famiglie e delle Forze armate, come ho già manifestato nella giornata di ieri in un messaggio inviato al capo di Stato maggiore della Difesa, generale Vincenzo Camporini. Voglio esprimere, inoltre, un sentimento di affettuosa vicinanza ai militari feriti nel corso dell'agguato, il primo caporalmaggiore Gianfranco Scirè e il caporale Cristina Buonacucina, rivolgendo loro un sincero augurio di pronta guarigione. In segno di lutto, invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

Desidero ringraziare lei, signor Presidente, e gli onorevoli colleghi per l'opportunità di poter riferire anche al Senato, come ho già fatto questa mattina alla Camera dei deputati, in ordine al gravissimo attentato avvenuto ieri mattina in località Mangan con la conseguente morte di due nostri soldati e il ferimento di altri due militari. In questa dolorosa circostanza voglio innanzitutto esprimere profondo e sincero cordoglio, non soltanto mio, ma, credo, di tutto il Governo e - se posso permettermi, signor Presidente - di tutta l'Assemblea, di tutto il Senato, come, questa mattina, di tutta la Camera, per la scomparsa di altri due militari, due militari, che hanno pagato con la vita la loro dedizione al dovere, il loro impegno, la loro consapevolezza di partecipare a una missione destinata a dare la pace a quello sfortunato territorio e più sicurezza

di Cuneo. Questo convoglio, formato non solo da militari italiani ma molto corposo (129 mezzi e 389 uomini) e destinato, oltre che a portare rinforzi, a sostituire i mezzi Lince che da molto tempo erano in quella base con quelli recentemente migliorati con una protezione aggiuntiva alla ralla ed altre protezioni, è stato

lo scoppio sotto uno dei mezzi Lince italiani. Era esattamente il quarto mezzo della colonna dopo i primi tre (quindi, era in realtà il settimo mezzo), con equipaggio afgano in ossequio alla nuova strategia che vede progressivamente sempre più impegnati i militari afgani, certo supportati da quelli del contingente internazionale. internazionale. In questo mezzo erano trasportati quattro guastatori del plotone ricognizione del Genio alpini, un plotone di ricognizione avanzato che aveva il compito di verificare il percorso e l'esistenza

a seguito dell'attentato sono deceduti due giovani alpini: il sergente Massimiliano Ramadù, di 33 anni, comandante del mezzo, nato a Velletri l'8 febbraio 1977, coniugato, e il caporalmaggiore Luigi Pascazio, di 25 anni, conduttore del mezzo, nato a Grumo Appula, in provincia di Bari, il 23 novembre 1985.

dell'aviazione americana, e da lì i medici hanno deciso di trasportarla nella base americana di Ramstein, in Germania. Noi non ci siamo opposti,

Signor Presidente, mentre ribadisco che restiamo in attesa delle notizie da Ramstein per la giovane ferita, possiamo sin d'ora dire che che è molto profonda la commozione ed è sincero il dolore per la perdita dei due giovani alpini. È una commozione vera che non riguarda solo noi, ma la stragrande maggioranza della nostra comunità nazionale che si stringe attorno al dolore dei familiari, che è vicina alle Forze armate, che sente come perdita grave e irreparabile la perdita di due ragazzi che hanno dato - lo ripeto - la vita per assolvere a un compito a cui li ha destinati la loro scelta di servire in armi l'Italia, ma anche la scelta della politica di contribuire a livello internazionale a una maggiore sicurezza e pace nel mondo e a un minore pericolo derivante dal terrorismo. Si è trattato nuovamente di un attentato compiuto con un ordigno cosiddetto improvvisato (IED), in questo caso di altissimo potenziale. Altre volte il Lince, il mezzo

all'aumento dell'efficienza dei mezzi difensivi corrisponde spesso un'accresciuta potenzialità della minaccia e dell'offesa: è una gara. Chi, come gara. Chi, come noi, sa che non siamo in guerra non può e non vuole mettere in campo i criteri, gli strumenti e le potenzialità che invece sono consentite in una guerra, e deve soprattutto badare a svolgere il proprio compito anche con l'uso della forza giusta, mettendo in campo tutte le difese possibili; a ciò però fra riscontro un aumento della potenzialità dell'offesa. In questo contesto credo che sia assolutamente necessario e inderogabile considerare prioritario il continuo aggiornamento e la continua ricerca di tutti i mezzi di protezione e di sicurezza di cui deve e può essere dotato essere dotato il nostro contingente. Nonostante il momento drammatico, sono in condizione di dirvi che finora nulla è stato lasciato al caso, e che noi siamo nella condizione di poter dire che quello che la politica (con la P maiuscola) poteva fare per mettere in condizione di massima sicurezza possibile (che non basta mai) i nostri soldati è stato fatto; ma non bisogna È per questo che oggi alla Camera mi sono permesso di dire che è lecito riflettere - io mi interrogo tutti i giorni al riguardo - se il gioco valga la candela. Tutti i giorni mi chiedo se i sacrifici che i nostri ragazzi fino a lasciare in quelle terre lontane addirittura il bene più prezioso, che è la vita, siano un gioco a cui valga la pena partecipare. il Governo, io, voi con il vostro voto al rifinanziamento delle missioni abbiamo dato è che il compito è così importante da consentire di chiedere questo enorme sacrificio ai soldati, che sono assolutamente consapevoli di ciò: negli incontri che ho avuto con loro ho visto la consapevolezza del rischio, ma anche la consapevolezza della necessità del loro impegno. Per questo, il nostro livello di gratitudine è ancora più alto e più importante.

Sono fermamente convinto della bontà delle nostre scelte, ma di una cosa - l'ho detto alla Camera e lo ribadisco - non si può discutere: la necessità che, una volta scelta la via della partecipazione alle missioni internazionali, non sia lesinata alcuna risorsa affinché i nostri soldati possano godere della massima protezione possibile e dei migliori mezzi di sicurezza esistenti

Peraltro, ha già terminato il periodo di addestramento (oltre che - prima - di approvvigionamento) un altro mezzo che si chiama Freccia. Ne abbiamo parlato in altre occasioni: si tratta di un mezzo un po' meno veloce e più voluminoso, ma che garantisce in determinate circostanze una sicurezza assai maggiore di quella del Lince, che pure continuerà ad essere utilizzato per gli usi tattici che i militari riterranno opportuni e necessari. Una domanda che ci siamo posti, che la stampa si è posta, che qualche politico si è posto è se l'attentato fosse diretto a colpire i soldati italiani. La risposta, purtroppo, viene dai fatti: nella stessa giornata un altro attentato ha colpito un soldato americano; questa mattina a Kabul c'è stato un altro attentato con molte perdite di vite umane; la colonna non era composta solo da italiani. La risposta dunque è molto semplice: l'attacco era rivolto alla missione internazionale, al contingente internazionale. Perché vi è una recrudescenza in questo periodo? Innanzitutto, perché è finito l'inverno, e noi sappiamo che questa questa attività è ciclica. Non bisogna poi dimenticare che vi è una volontà destabilizzante crescente. Ma il motivo che noi riteniamo più importante di tutti è connesso all'avvio del piano McChrystal, del piano McChrystal, che prevede un maggior controllo del territorio, anche attraverso - proprio quello che stavamo facendo - l'arrivo di rinforzi nelle basi avanzate. È vero che larga parte del territorio fino a ieri è stata assolutamente

né cercando di fermare, attraverso attentati terroristici, la colonna. Vi siete chiesti - questo non l'ho riferito questa mattina alla Camera - quale fosse lo scopo di questo attentato? Normalmente noi portiamo rinforzi di materiale e di uomini. Lo scopo dei terroristi doveva essere quello di bloccare l'arrivo di questi rinforzi. Non ci hanno neanche provato.

con l'arma vile, subdola e vigliacca del terrorismo non per fermare l'azione militare, che pure è improntata al massimo rispetto dei compiti che ci hanno affidato gli organismi internazionali, ma per cercare di minare la volontà dei popoli e dei Governi che fanno parte di quella missione nell'intento di bloccare il terrorismo.

in realtà non vogliono far altro che strizzare l'occhio ad un pacifismo unilaterale, che in Italia c'è sempre stato, per una posizione che posso anche comprendere e rispettare, ma mai condividere: mai condividere! Il Il piano McChrystal, cui è ispirata la nostra azione, ha l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e di conquistare il cuore e le menti degli afgani attraverso una maggiore azione di di ricostruzione, una maggiore vicinanza, una forte sollecitazione al Governo afgano a far crescere il rispetto dei diritti umani in quella terra. Questo dà molto fastidio ai terroristi, perché è l'opposto di ciò che vorrebbero. Noi italiani questa strategia l'abbiamo sempre rivendicata, l'abbiamo sempre pensata, oltre che, nel nostro piccolo, cercato di predicare. Oggi che diventa la strategia della missione internazionale, dobbiamo supportarla nel migliore dei modi e far sì che possa essere foriera di un risultato positivo secondo i tempi che ci siamo dati: 2011, inizio del rientro dei soldati aggiuntivi inviati; 2013, affidamento della questione afgana al legittimo Governo afgano, alla polizia afgana, alle forze armate afgane, cui progressivamente stiamo già dando un ruolo maggiore. Nessuno s'immagina che da qui al 2013 vengano meno le minacce in Afghanistan, ma possiamo ragionevolmente immaginare, e volere, che entro quella data la afganizzazione della questione sia stata compiuta, e tocchi al legittimo Governo afgano e alle sue forze militari e di polizia affrontare e contrastare il terrorismo, così come il traffico di droga e la criminalità organizzata.

nella consapevolezza della sua valenza, per la stabilizzazione dell'Afghanistan e per la lotta al terrorismo internazionale. Un impegno - voglio leggere le parole stesse che ho usato alla Camera che non sarà certo messo in discussione da questo vile attentato. Personalmente ho incontrato i militari in Afghanistan più volte, e ho visto che questo è anche il loro sentimento, quello di far sì che non sia vano l'impegno di chi si è alternato in quella terra per ridare già risultati concreti: la la democrazia che avanza, le scuole che si aprono, le donne che cominciano con molta fatica ad avere diritti; l'impegno per arrivare ad una situazione ancora migliore; ma, soprattutto, l'impegno - lo ripeto perché siano minori i pericoli derivanti dal terrorismo nelle nostre case, nelle nostre città, nelle nostre Nazioni. Concludo, dando atto del meritorio comportamento dei nostri militari in Afghanistan, dove operano senza dubbio in un contesto difficile e complesso. Ma lo stanno facendo con grande equilibrio, competenza e professionalità dicevo prima, dalla convinzione dell'utilità del loro ruolo. Questa sicurezza la garantiscono migliaia di uomini che hanno scelto tale strada. Consentitemi di dirlo, e non mi si accusi di chissà quale spirito militaresco. Consentitemi di dire che oggi l'apprezzamento che essi riscuotono in ogni parte del mondo fa sì che, accanto alle grandi eccellenze che l'Italia ha sempre vantato (l'arte, la cultura, più recentemente la moda, il *design*),

che gli organismi internazionali affidano loro. Credo che oggi i nostri ragazzi e le nostre ragazze con le stellette siano veramente una eccellenza che ci deve e ci può far inorgoglire. Ed alle ragazze con le stellette, alle donne, oggi che oggi che una di loro, per la prima volta, viene ferita seriamente, credo si voglia tutti insieme riconoscere un *plus* di solidarietà, di gratitudine, di vicinanza, perché hanno dimostrato, al pari dei loro colleghi uomini, di essere in grado di svolgere al meglio il loro compito. A loro, credo, un *plus* di sicurezza e di gratitudine deve e può essere riconosciuto. Voglio concludere leggendo l'ultima parte perché sia chiaro, e mi rivolgo certamente agli infami, vigliacchi aggressori che hanno colpito anche stavolta nella maniera più subdola, ma anche alle orecchie che hanno qui in Italia e che riferiscono ogni dettaglio di quello che la politica e le istituzioni dicono e fanno in ragione di quello che avviene in Afghanistan. Ed ho l'orgoglio di dire che la politica con la "P" maiuscola - quella che si è manifestata con il voto unanime di rifinanziamento delle missioni internazionali, una politica orgogliosa in questo caso della propria unità al di là degli schieramenti - e le le istituzioni mandano a dire (e se ci sono orecchie che ascoltano, e ce ne sono, riferiscano) che rimane più che mai saldo l'intendimento del Parlamento e del Governo di mantenere l'impegno italiano per la stabilizzazione dell'Afghanistan. Ribadisco, pertanto, che anche questo drammatico episodio avrà come effetto il rafforzamento del nostro convincimento sulla presenza italiana in Afghanistan e sul nostro apporto alla missione ISAF. La nostra vicinanza ai soldati italiani è più forte che mai, il nostro convincimento del loro ruolo è più sicuro e doveroso che mai. *(Prolungati

E se ieri, signor Ministro, era il giorno del lutto, del cordoglio, della sofferenza... *(Vivaci

se ieri era il giorno del lutto, del cordoglio, della sofferenza e del silenzio, oggi è il giorno della parola, della riflessione politica e anche della critica, perché da questa Aula non deve uscire solo un momento di dolore, assolutamente doveroso, ma non sufficiente, perché rivolto soltanto al passato, ma deve sortire anche un progetto che guardi al futuro. Ieri sono morti il sergente Massimiliano Ramadù ed il caporalmaggiore Luigi Pascazio. Sono morti ad Herat, mentre stavano portando avanti una missione che il Governo aveva loro detto essere di pace, mentre facevano ricostruzione e aiuto alla popolazione afghana che il Governo gli aveva garantito esserci grata e riconoscente, mentre onoravano la nostra Patria e la nostra Costituzione, che il Governo gli aveva assicurato essere una Costituzione pacifista, che all'articolo 11 rinnega la guerra come strumento d'offesa. Colleghi, questi giovani non si erano sbagliati indossando la divisa per servire l'Italia, rischiando la loro vita per la sicurezza internazionale e per la difesa del nostro Paese. E a loro va il pensiero di gratitudine, di orgoglio, di amore dell'Italia dei Valori e dell'Italia intera. Chi si era sbagliato e chi sta sbagliando anche adesso, purtroppo, è il Governo. Ho sentito dalle sue parole, signor Ministro, che «il gioco vale la candela»;

anche astenendoci sul finanziamento delle missioni e votando contro l'articolo che regola nello specifico la missione afgana, oggi ancor di più non possiamo tacere. Le famiglie dei caduti ci chiedono di fare in modo che la tragedia dei loro figli non sia inutile. A noi ciò che fa più paura è che invece l'inutilità sarà assicurata se non avverrà un mutamento di paradigma nella politica estera del Governo.

o di che mezzi rifornire, ma nella strategia generale che si intende perseguire, in Afghanistan come in altri teatri, per contribuire lealmente agli sforzi della comunità internazionale e, allo stesso tempo, valorizzare quello che il nostro Paese sa e può fare meglio. Se non si passerà cioè da un gioco al rialzo militare ad un progetto di riconversione civile cominciando a ridurre le spese della Difesa, che anche il decreto incentivi aumenta, investendo in piattaforme militari multifunzione (nonostante fosse una norma presentata per aiutare le fasce più deboli del nostro Paese); se non cominciamo ad aumentare le risorse del Ministero degli esteri, rivalutando una cooperazione allo sviluppo ormai scaduta in qualità e quantità dell'impegno; se non si arriverà ad ammettere che la sicurezza in Afghanistan non è né perfetta né perfettibile in uno scenario ormai completamente mutato dall'inizio della missione; se non si esternerà finalmente la volontà di uscire dal "pasticcio" afgano con una seria e condivisa *exit* *strategy* che non mortifichi i partner NATO ed europei, ma nemmeno le vite dei nostri soldati, se non riusciamo in tutto ciò, l'Italia dei Valori si ritroverà ancora una volta a fare la Cassandra in un Parlamento di ciechi e di sordi. Noi non vogliamo essere premonitori di tragedie annunciate, vogliamo contribuire alla politica estera italiana e alla sicurezza internazionale, ma solo partendo da una onestà di fondo, che finora il Ministro della difesa non ha dimostrato,

colleghi! Di guerra si muore, di disorganizzazione nella gestione di questa si muore, di mancanza di onestà intellettuale nella valutazione del presente e del futuro.Quello che chiediamo oggi, pur sapendo di essere futuro.Quello che chiediamo oggi, pur sapendo di essere i soli a farlo, è la stessa cosa che ripetiamo da più di un anno: ci si impegni quando il nostro sforzo è legittimo, costituzionale e utile, ma si convertano i nostri sforzi quando giornate come quella di ieri testimoniano tristemente all'Italia un errore macrostrategico che i nostri più valorosi cittadini non devono pagare. Cambiamo pagina, solo così la commemorazione di oggi avrà un senso.

profondo convincimento e con intima solidarietà, alle sue parole di cordoglio per la scomparsa del sergente Massimiliano Ramadù e del caporalmaggiore Luigi Pascazio, così come alle parole di augurio di pronta guarigione per Cristina Buonacucina e Gianfranco Scirè. non è la prima volta che in quest'Aula siamo chiamati ad esprimere il dolore per la perdita di nostri militari impegnati in missioni internazionali di pace, e non è la prima volta che le istituzioni del nostro Paese sono chiamate a dimostrare, al di là della consuetudine e della formalità, l'intima e sincera solidarietà umana, politica e istituzionale a tutti i militari che in questo momento si trovano impegnati in Afghanistan, così come in tutte le missioni internazionali che vedono il nostro Paese in prima fila. Io credo, signor Presidente, signor Ministro, che il modo migliore per essere utili in questo momento, al di là delle parole di circostanza, di circostanza, e per essere sinceramente vicini ai nostri militari sia dire con chiarezza due cose. La prima che noi ci sentiamo di dire, senza infingimenti, con determinazione e con responsabilità, è che riteniamo che sia giusto stare lì, che sia giusto stare lì, continuando l'impegno internazionale del nostro Paese e rafforzando in termini di risorse umane, economiche e militari lo sforzo che il nostro Paese sta facendo in Afghanistan, perché è uno sforzo utile. infatti, siamo lì per formare il personale della polizia, per far crescere una nuova società civile afgana, con istituzioni forti che siano in condizione di governare quel Paese, un Paese difficile, in uno scenario difficile,

per farlo - al modo di migliorare le condizioni e l'efficienza del nostro impegno in Afghanistan e in tutte le missioni internazionali di pace. Questo è il tema di cui ci dobbiamo occupare e non la sterile, stucchevole e di pessimo gusto disputa sul ritiro o meno dei nostri militari in questo momento. Noi condividiamo, signor Ministro, la dichiarazione che lei ha fatto in quest'Aula, relativa al fatto che l'ipotesi di un disimpegno possa essere in qualche modo interpretata, da chi barbaramente attenta alla vita dei nostri militari in quel Paese, come una istigazione o un incentivo. Noi riteniamo che questo sia profondamente vero e per queste ragioni, oltre ad associarci al dolore dei familiari e a solidarizzare, «senza se e senza ma», con i nostri militari impegnati in quel territorio, le diciamo che non verrà mai meno il sostegno del nostro Gruppo parlamentare alle missioni e a ciò che il Governo intenderà fare nell'interesse del Paese in quello scenario difficile che tutti noi abbiamo voluto cambiare insieme. finestra") *(LNP)*. Signor Ministro, colleghi, l'attentato che è costato la vita a due militari del Genio guastatori alpini uccisi ieri mattina nella provincia di Herat ci ricorda una volta di più le difficoltà ed i grandi costi umani della nostra missione in Afghanistan. Quanto accaduto costituisce per me un motivo di particolare dolore, avendo presenziato, unitamente al Ministro della difesa, al sottosegretario Crosetto e ad alcuni colleghi, come la senatrice Bonfrisco e il mio collega di Gruppo Vaccari, alla sfilata degli alpini di una settimana fa Mentre ci inchiniamo davanti al sacrificio dei nostri ragazzi ed al dolore delle loro famiglie, vogliamo sottolineare in questa triste occasione come in Afghanistan i soldati del nostro Paese non siano soli. La Lega Nord li sosterrà sempre. Operiamo infatti nel contesto di una grande alleanza occidentale che è lì con l'autorizzazione delle Nazioni Unite per sradicare il terrorismo internazionale e soprattutto per restituire la speranza di un futuro migliore ad un popolo, quello afgano, Il carattere condiviso e non meramente nazionale dell'impresa spiega la posizione di responsabilità assunta dal nostro partito, che, che, pur richiamando le dichiarazioni rese in passato, conferma la necessità assoluta di rimanere fedeli agli impegni presi con il Governo e con i Paesi alleati in merito a questa che, lo sottolineo, è Commentando a caldo questa notizia, il ministro Bossi ha affermato che lasciare l'Afghanistan adesso equivarrebbe ad una fuga dagli esiti imprevedibili, sia nei rapporti con i nostri alleati, che non riuscirebbero a capirne il motivo,

tanto più che questo impegno non ha comportato soltanto l'uso delle armi, ma anche interventi importanti sulle infrastrutture e sui servizi di base che sono stati messi a disposizione del popolo afgano. Oggi dobbiamo ricordarci che in quel martoriato Paese ci sono più strade, ponti, scuole ed ospedali di quanti non ne esistessero quando c'erano i talebani.

che unanimemente sembrano privilegiare il 2013 come data per il ritiro di tutti i contingenti.

delle famiglie, ma anche esprimere un augurio immenso ai due militari feriti, soprattutto alla ragazza, per una pronta guarigione, dicendo loro che la Lega Nord non sarà mai lontana dai nostri militari.

signor Ministro, onorevoli colleghi, il Partito Democratico, come tutti gli italiani, esprime grande cordoglio e forte vicinanza alle famiglie dei caduti, invia un affettuoso saluto ai feriti, con l'auspicio di una loro pronta guarigione ed in particolare, dopo le sue parole, signor Ministro, al caporale che in questo momento è sottoposto ad intervento chirurgico. I nostri soldati ancora una volta hanno dimostrato la loro dedizione ad un difficile compito fino ad arrivare, purtroppo, all'estremo sacrificio. Non è questo certamente il momento della retorica, ma dobbiamo rimanere e guardare a questa situazione da un punto di vista oggettivo per poter dare risposte a tutti gli interrogativi che in questi giorni abbiamo sentito rivolgerci dall'opinione pubblica. Questi interrogativi devono avere una risposta che deve partire dalle ragioni dell'impegno della comunità internazionale in Afghanistan. Va ricordato innanzitutto che sono 42 le Nazioni che operano in quel teatro, ma soprattutto che questa presenza è stata decisa nel 2001 e negli anni successivi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, un'organizzazione internazionale prevista nell'articolo 11 della Costituzione, alla quale naturalmente l'Italia, come tante altre Nazioni, ha ceduto e cede parte della propria sovranità internazionale. L'operazione in Afghanistan ha raggiunto dei risultati positivi in questi anni e forse sarebbe ingeneroso non riconoscerlo oggi, anche per ricordare l'impegno di quei soldati che purtroppo hanno perso la vita. Nel 2005 è stato eletto democraticamente il Parlamento afgano: erano 30 anni che questo non accadeva. È stata avviata una riforma della giustizia nella quale l'Italia ha avuto un ruolo importante; si stanno costruendo le forze di sicurezza nazionali, in un Paese che prima era diviso tra una moltitudine di poteri locali; l'istruzione dei giovani, che nel regime talebano non potevano accedere alla cultura o alla crescita sociale, è diventato un obiettivo primario; è stata anche avviata la ricostruzione delle istituzioni democratiche e delle infrastrutture. Certo, si tratta di riforme realizzate o avviate con grande difficoltà, ma che sarebbero state impensabili senza la presenza della comunità internazionale. Purtroppo, l'aumento degli incidenti indica che il processo di stabilizzazione non è ancora concluso. Non si tratta di disconoscere a mio modo di vedere le ragioni che sono alla base della presenza in Afghanistan. Un abbandono dell'Afghanistan in questo momento da parte della comunità internazionale farebbe probabilmente crollare il Paese nelle stesse condizioni da cui la stessa comunità vuole e voleva trarlo. Si tratta però di verificare, insieme alle Nazioni partecipanti e agli organismi internazionali che hanno promosso questo impegno, se sia opportuno correggere ed in quale misura la missione se la comunità internazionale non debba accentuare gli sforzi a favore di un processo sociale ed economico del Paese che consenta di conquistare i corpi e le menti della popolazione afgana, che è la condizione indispensabile per ottenere un risultato positivo. In tale contesto, le innovazioni apportate dal presidente Obama alla strategia dell'operazione in Afghanistan devono essere un riferimento costante per il contributo italiano alla missione. La maggiore attenzione verso la popolazione e la ricostruzione, che è stata sollecitata dal Presidente, non può non essere sostenuta con forza dall'Italia, visto che coincide con la linea politica da sempre seguita dalla nostra Nazione nelle missioni di stabilizzazione. E così la necessità di evitare le vittime civili, anch'essa richiamata dal presidente Obama, non può non vederci convinti assertori, considerate le conseguenze altamente negative che i danni collaterali, purtroppo, determinano nella ricerca del consenso della popolazione. Ed ancora, lei ne ha parlato, signor Ministro, l'afganizzazione della crisi, attraverso la realizzazione della più rapida possibile delle condizioni per la cessione della responsabilità al Governo afgano, deve trovare anche in questo caso l'Italia tra i Paesi più coinvolti. Infine, il nuovo processo di riconciliazione nazionale con la parte moderata dell'insorgenza è un passaggio cruciale per superare la violenta contrapposizione interna al Paese, che vanifica gli sforzi di pacificazione. Anche in questo caso, l'Italia può e deve dare un contributo che nasce dalla sua moderazione e dal suo ruolo di garanzia.

onorare la loro memoria continuando ad operare con equilibrio e professionalità in quel teatro, predisponendo la sua attività predisponendo la sua attività politica in maniera che le riflessioni che oggi stiamo facendo possano essere domani il viatico non solo per il contingente italiano, ma per il contingente di tutto l'ISAF. Chiedo

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo apprezzato molto la sua relazione, che ha evidenziato, con puntualità con estrema chiarezza, la missione dei nostri soldati, che onorano il Paese con il loro sacrificio, in un costante orgoglio che rappresenta il nostro Paese nei vari scenari internazionali. Ieri, nelle dolorose ore che hanno seguito la notizia dell'attentato in Afghanistan, quando ha preso corpo il reale contenuto della tragedia e si sono conosciuti i nomi e i volti delle vittime, tra le migliaia di dichiarazioni che si sono succedute - alcune anche abbastanza curiose - una merita senz'altro di essere ricordata. Consentitemi di leggerla: «È un dolore per ogni uomo con un cuore, per ogni uomo che crede nel sacrificio per la Patria, per ogni uomo che crede negli ideali, che dare un contributo piccolo o grande che sia possa servire a migliorare il mondo anche con la propria vita». Sono le nobili parole di Angelo Pascazio, il papà del caporalmaggiore Luigi,

e che, ciò nonostante, parla di sacrificio per la Patria, di ideali, della necessità di dare il proprio contributo per migliorare il mondo. È una lezione che ci ha dato questo papà. Sono parole che devono far riflettere tutti, specie quanti - probabilmente numerosi, ahimè - sull'onda delle emozioni, si sono fatti tentare dall'idea di far rientrare i nostri militari, creare polemiche, convincendosi dell'inutilità di una missione che sembra non portare benefìci. Ma non è così. Far rientrare oggi i nostri soldati o ridimensionare quantitativamente o qualitativamente il nostro impegno significherebbe davvero rendere vana la missione fin qui condotta e inutile il tributo di sangue che l'Italia ha finora versato in Afghanistan contro il terrorismo, in un processo di democrazia in un'area estremamente instabile. Mai come oggi bisogna invece mantenere gli impegni internazionali, assunti sulla base delle alleanze e del vincolo che abbiamo preso con il popolo afgano e con il mondo intero. Il contingente italiano - ricordiamolo - è in Afghanistan non per combattere ma per dare un contributo attivo ai necessari processi di democratizzazione dell'area e alle attività volte a migliorare le condizioni di una popolazione duramente provata da circa un trentennio di guerre e di situazioni connotate da alta instabilità e da altissima malavitosità, con un centro di smercio di droga mondiale. La presenza delle nostre truppe oggi è più che mai necessaria, per permettere la stabilizzazione e la pacificazione di una vasta area dell'Asia che comprende, oltre all'Afghanistan, altre regioni calde - penso per esempio al Pakistan, alla Thailandia in queste ore - e che rappresenta una delle principali sfide non solo della NATO, ma dell'intera comunità internazionale, nell'ambito della quale i nostri militari forniscono quotidianamente un contributo fondamentale. Sarebbe insensato ritirarsi proprio oggi,

e alla comunità internazionale le proprie scelte. L'Italia è orgogliosa dell'impegno dei suoi militari. È vicina in questo momento e sempre alle famiglie dei caduti, e continuerà ad impegnarsi per promuovere la pace fra le Nazioni. Questa missione, alla quale non possiamo né vogliamo sottrarci, rimane la certa volontà del Paese e delle sue Forze armate, anche in questo momento di grande dolore in cui l'Italia e il Popolo della Libertà onorano onorano il coraggio e il valore dei suoi giovani caduti: il sergente Massimiliano Ramadù e il caporalmaggiore Luigi Pascazio.

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 maggio. Il decreto-legge in materia di incentivi, già all'ordine del giorno dell'odierna seduta, si trova tuttora all'esame delle Commissioni competenti. Pertanto, subito dopo la lettura del calendario, la seduta dell'Aula sarà tolta per consentire il prosieguo dell'esame in sede referente e il conferimento del mandato ai relatori. La discussione da parte dell'Assemblea è quindi rinviata alla seduta antimeridiana di domani e il pomeriggio di oggi resta riservato ai lavori delle Commissioni. Il calendario della settimana corrente prevede inoltre - ove possibile in relazione all'andamento dei lavori - l'esame della ratifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia e il seguito del disegno di legge di riforma della professione forense. Nella seduta antimeridiana di giovedì 20 maggio avrà luogo, per la durata di 2 ore - dopo le ore 11 in relazione all'andamento dei lavori - il dibattito sul 40° anniversario dello Statuto dei lavoratori. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi. La prossima settimana, dal 25 al 27 maggio, è previsto 1'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge su sospensione temporanea demolizioni in Campania e stabilità finanziaria dell'area euro. Per il dibattito su quest'ultimo provvedimento è stato richiesto 1'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze. Nella seduta pomeridiana di martedì 25 maggio, la Presidenza ricorderà il 200° anniversario dell'indipendenza della Repubblica Argentina. Successivamente i rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire per 5 minuti ciascuno. Nella seduta pomeridiana di giovedì 27 maggio, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro del lavoro risponderà a interrogazioni a risposta immediata in tema di Cassa integrazione guadagni. In relazione alla festività di mercoledì 2 giugno, è stato stabilito che 1'Assemblea sarà convocata nel pomeriggio di lunedì 31 maggio e la mattina di martedì 1° giugno per la discussione degli argomenti che saranno definiti dalla prossima Conferenza dei Capigruppo, da convocare nella giornata di martedì 25 maggio. Il Parlamento in seduta comune sarà convocato giovedì 1° luglio, alle ore 9, per l'elezione di 8 componenti del Consiglio superiore della magistratura. La chiama inizierà dagli onorevoli senatori.

contrasti riguardo all'organizzazione dei lavori di queste tre Commissioni e, soprattutto, delle sovrapposizioni anche con sedute notturne. In particolare, anche questa sera è prevista una sovrapposizione fra la Commissione giustizia e la Commissione antimafia.

importante, anche perché alla Marcia per la pace di Assisi erano presenti centinaia e centinaia di giovani, centinaia di persone impegnate quotidianamente nella lotta

«La guerra che stiamo conducendo in Afghanistan ci ha restituito questa mattina altri corpi straziati di soldati italiani. Altri morti, altri feriti, altro dolore, altro sangue che costringono tutti a riaprire gli occhi su questa tragedia. La morte, il dolore e il sangue scorrono tutti i giorni in Afghanistan (...). Di questa guerra gli italiani non sanno quasi nulla. Qui in Italia, nelle retrovie della guerra, siamo sottoposti al ferreo regime della censura. Qui (come in nessun altro Paese al mondo), dall'11 settembre 2001 è persino vietato chiamare le cose con il loro nome. L'espressione "guerra in Afghanistan" è bandita. Ma tutto questo non ci aiuta a capire cosa dobbiamo fare. "Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge. Qualsiasi appello all'odio nazionale razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge Il dolore dei familiari dei soldati uccisi e l'angoscia di quelli feriti gravemente è anche il nostro. È un dolore forte, che ci deve spingere a fare qualcosa in più per fermare e non continuare a combattere questa guerra. I nostri giovani soldati muoiono, perché il Governo continua a scaricare sui militari il compito di risolvere un problema che i militari non hanno nessuna possibilità di risolvere.